Nella seduta di domani, con inizio alle ore 11,15, il Ministro dell’interno renderà un’informativa sulla vicenda della nave Aquarius. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Martedì 19 giugno, a partire dalle ore 11 e senza orario di chiusura, sarà discusso il Documento di economia e finanza 2018. Il calendario della settimana prevede inoltre la discussione del decreto-legge recante ulteriori misure a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. L’esame del provvedimento, ove non concluso, potrà eventualmente proseguire nella settimana dal 26 al 28 giugno.

Il calendario potrà essere integrato con un’informativa del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali sugli incidenti nei luoghi di lavoro. Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 21 giugno, alle ore 14,30, per l’elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori. Comunico infine che i Gruppi dovranno far pervenire alla Presidenza le designazioni dei propri componenti nelle Commissioni permanenti e nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari entro le ore 20 di lunedì 18 giugno.

colleghe senatrici e colleghi senatori, a nome del Gruppo Partito Democratico, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, del Regolamento del Senato, avanzo la proposta di modifica del calendario per introdurre e calendarizzare la mozione proposta dal Partito Democratico sul reddito di inclusione. Il nostro obiettivo è di discutere nelle Aule parlamentari, non su Facebook e non inseguendo dichiarazioni a mezzo stampa, di un problema problema sentito da molti concittadini in condizioni di bisogno, dagli enti locali e dal terzo settore, per dare certezza su un tema così importante. Da cento giorni il Parlamento è bloccato, le Commissioni non si sono ancora costituite perché dobbiamo aspettare trattative più o meno trasparenti su ben altro. Potevamo discutere del decreto-legge terremoto già questa settimana; si è deciso di farlo la prossima. Chiediamo di discutere in Assemblea di provvedimenti e problemi urgenti e importanti. Perché il reddito di inclusione? Perché dal primo luglio questa misura introdotta nella scorsa legislatura diventerà pienamente universale, grazie alle risorse stanziate nell’ultima legge di bilancio - finalmente, checché se ne dica - e anche nel programma di Governo, nonostante ancora si lamenti, restando un po’ indietro rispetto al dibattito degli anni Novanta,

i Governi del Partito Democratico hanno inserito una misura unica di contrasto alla povertà: il reddito di inclusione. Quando siamo arrivati al Governo, in questo Paese si spendevano 40 milioni di euro sperimentali per il contrasto alla povertà;

Dobbiamo dare una risposta chiara alle famiglie, alle persone coinvolte, sulle risorse che ci sono a finanziare il reddito di inclusione. Si sente parlare, nei mezzi di informazione, di proposte mirabolanti di contrasto alla povertà, senza coperture, senza certezza sui tempi. Alcuni esponenti della maggioranza e del Governo parlano di rinviare l’introduzione del reddito di cittadinanza di qualche anno perché prima bisogna riorganizzare i centri per l’impiego.

In tutti i sistemi di welfare ci sono due strumenti per dare garanzia del reddito a chi è in condizioni di bisogno: uno strumento più assicurativo, legato alla storia contributiva, e uno assistenziale, sottoposto alla prova dei mezzi. Finalmente, come dicevo, nella scorsa legislatura anche lo stato sociale italiano si è dotato del secondo, con risorse certe e a regime. Nel dibattito sui giornali e sui social di questi giorni si continua a fare confusione tra gli strumenti: quelli legati alla storia contributiva e quelli sottoposti alla prova dei mezzi. Per dare certezza non solo alle famiglie in condizioni di bisogno ma ai Comuni, al terzo settore, alle associazioni che per troppi anni sono state lasciate sole a combattere in trincea contro la marginalità sociale e le condizioni di povertà, dal Parlamento e dal Governo devono arrivare parole chiare sulle

non era soltanto un trasferimento monetario, ma anche uno strumento di attivazione sociale, ancor prima che lavorativa, e devono esserci, non per niente, risorse certe non solo per i centri per l’impiego ma anche per i servizi sociali, per il terzo settore e per chi deve far vivere i servizi, accompagnando le famiglie in condizioni di fragilità sociale. su Facebook né in altri luoghi, devono arrivare parole chiare e certe sulle risorse e sugli strumenti che si intende mettere in campo per il contrasto alla povertà. Ci sono due modi per essere vicini ai cittadini: uno è prenderli in giro con mirabolanti proposte elettoralistiche; l’altro è guardarli negli occhi e dire con chiarezza quali sono gli strumenti che li accompagneranno, soprattutto quando si trovano condizioni di bisogno e fragilità. Il Partito Democratico, nella scorsa legislatura, ha scelto il secondo approccio, chiediamo alla maggioranza e al Governo di dirci qual è il loro.

che questa Assemblea esamini al più presto questa mozione. La tutela dei diritti umani - lei, Presidente, me lo insegna - rappresenta uno degli elementi fondanti dell’ordinamento nazionale e anche del rapporto tra

in proposito, perché - torno a ripetere - sono ben due legislature che questa Commissione è stata istituita al Senato e credo che oggi ancora più

Signor Presidente, anche noi chiediamo l’inseri- mento di una mozione, che gli uffici stanno per ricevere, affinché il Governo comunichi con la massima tempestività le modalità e i tempi con i quali intende intervenire per prevenire l’aumento dell’IVA con il passaggio al nuovo anno, sulla base delle clausole di salvaguardia. clausole di salvaguardia. Sappiamo bene della turbolenza dei mercati finanziari di questi tempi, dell’incertezza che crea negli investitori in generale e in particolare negli investitori finanziari una situazione per la quale

cosa è dire che lo si farà e un’altra cosa è definirne i tempi e i modi, che potrebbero davvero rassicurare gli investitori e dare un orizzonte più chiaro e sereno alla nostra economia e agli investitori che puntano sui titoli di

Signor Presidente, chiedo l’attenzione, oltre che dell’Aula, specificatamente della senatrice De Petris. La senatrice De Petris ha proposto la calendarizzazione della mozione per la costituzione della Commissione dei diritti umani. tale proposta è stata sottoscritta trasversalmente da praticamente tutti i Gruppi presenti in quest’Aula e condividendo la sua iniziativa, sono a proporre alla senatrice De Petris

senatrice De Petris.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, domenica 3 giugno è scomparso a Udine, all’età di novantacinque anni, il senatore Mario Toros, una della personalità politico-istituzionali più significative del Dopoguerra di tutto il Friuli-Venezia Giulia e punto di riferimento per molti esponenti politici della mia Regione. A lui alla sua azione politico-amministrativa il Friuli-Venezia Giulia deve molto, nel contesto degli anni difficili della ricostruzione postbellica e del post-terremoto; anni in cui la Regione è riuscita a percorrere strade nuove e a raggiungere obiettivi ambiziosi, per taluni definiti addirittura insperati. Mario Toros nasce in una famiglia contadina di Feletto Umberto. Avendo frequentato le scuole professionali, ha una formazione da autodidatta. Mario Toros aderisce ai gruppi di Azione Cattolica e delle ACLI. All’età di quattordici anni entra come operaio nelle fonderie Bertoli di Udine: un’esperienza - ripeteva Da antifascista Toros partecipò alla Resistenza, combattendo nella Brigata partigiana Osoppo Friuli. Nel 1950 fu tra i fondatori della CISL e molto presto aderì alla Democrazia Cristiana. Aclista e cattolico e cattolico convinto, nel Friuli devastato dalla guerra assurge a figura politica di riferimento, dapprima come consigliere comunale a Tavagnacco e, poi, a Manzano. Eletto nel primo Consiglio provinciale di Udine, ricopre il ruolo di assessore. Nel 1958

carisma, sensibilità e capacità pazzesca di arrivare al cuore delle persone, come, all’indomani della scomparsa, ha detto di lui uno dei suoi cinque nipoti. Nel corso della lunga esperienza romana fu Sottosegretario al lavoro con tre diversi Presidenti del Consiglio e più volte Ministro della Repubblica, prima alle Regioni e, poi, al lavoro e alla previdenza sociale. Toros si spese molto per l’autonomia e la specialità della Regione Friuli-Venezia Giulia. Fu fedele interprete dell’identità culturale della propria terra, dalle radici plurime. Con lui scompare un testimone nobile e illuminato di un tempo difficile. Il presente e il passato sono dei mezzi - dirà il fine è il futuro. È questo che piace nel ricordare Mario Toros. Penso sia determinante non lasciare nell’oblio chi ci ha preceduti, in particolare quando una persona si identifica con la propria comunità e ne diventa portavoce per eccellenza,

non solo del Friuli, ma - credo - del nostro Paese. Mario Toros è stato un importante sindacalista, un senatore, un deputato e più volte Ministro e Sottosegretario del lavoro.

Presidente, vorrei associar- mi anch’io al ricordo dei colleghi. Mario Toros è stato uno degli interpreti più significativi della corrente sindacale della Democrazia cristiana che faceva capo a Carlo DonatCattin, onorando a più riprese il Senato e il Parlamento. È stato un grande Ministro del lavoro e una delle personalità più significative per il rapporto con il territorio, che ha sempre coltivato, e per tutte

Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 13 giugno